Signora Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori a nome del Gruppo di Forza Italia, cogliendo anche l'occasione della presenza dei rappresentanti del Ministero degli affari esteri e per chiedere alla Presidenza, anche previa eventuale Conferenza dei Capigruppo, di calendarizzare per i prossimi giorni un intervento in Aula del Governo,

le cronache e anche le attività parlamentari. Il Senato ha ben titolo per chiedere un intervento preventivo del Governo, in quanto è una sede dove la questione è stata ampiamente discussa ed è l'unica sede dove vi è stato un atto di indirizzo, peraltro assunto all'unanimità

artefici di una discussione che ha portato, caso abbastanza raro, all'approvazione di un documento unanime, dal quale poi è scaturita, non a caso, tutta l'azione riguardante la regolamentazione delle ONG e il dibattito che si sta svolgendo.

di questo accordo Sophia. Leggo anche che l'Italia, cosa che apprezzo, ha assunto un atteggiamento più vigoroso rispetto al passato, chiedendo la revisione di questi interventi e dell'operazione Triton. Insomma,

forse a livello di Presidenza del Consiglio o comunque dei Ministeri che gestiscono questi *dossier*, che sono diversi: gli esteri, certamente; l'interno, certamente; la difesa per i suoi aspetti, perché le operazioni sono fatte

però mi paiono riunioni ancora più decisive, visto il contenuto. Avendo il Senato approvato all'unanimità un documento di indirizzo, avere poi in Aula un confronto preventivo con il Governo potrebbe rafforzare - lo dico anche ai Sottosegretari - il mandato del Governo della Repubblica italiana, che potrebbe

il punto in cui c'è la massima chiarezza, da parte del Governo e da parte dei parlamentari, rispetto al popolo italiano. Recentemente, rispetto all'operazione Triton,

invece, che questo discendeva dalla richiesta dell'Italia che tutte le navi, qualunque bandiera battessero, portassero i rifugiati o gli immigrati irregolari in Italia. Credo che questa sia una responsabilità enorme del Governo italiano, nelle persone del presidente del Consiglio Renzi, dell'allora ministro degli affari esteri Gentiloni e del ministro dell'interno Alfano.

il trasporto degli emigrati clandestini dalla Libia in Italia, al punto che, sotto l'egida dell'ONU, si sarebbe potuti andare ad affondare le barche anche sul suolo libico, ed è diventata, di fatto, l'ennesima ambulanza, taxi o come diavolo volete chiamarla, per portare gli emigranti in Italia. A questo punto, il Governo abbia un mandato parlamentare: l'operazione Sophia, per come era stata impostata, si fondava su presupposti di difesa e non di continuo soccorso: intento originario, per far sì che, con l'accordo dell'ONU e finalmente anche della Libia, non si continui a trasformare questo Stretto in un ponte,

di discutere, prima della scadenza della missione Sophia, un atto di origine parlamentare, così come è stato fatto, in maniera assolutamente costruttiva e produttiva, dalla Commissione difesa del Senato.

dell'Alleanza atlantica, possono essere installate anche a bordo di altre Nazioni NATO che non possiedono armi nucleari.

dovremmo meditare se il nostro modello di difesa possa veramente concepire qualcosa del genere: mettere due bombe della potenza pari a venti volte quella di Hiroshima a bordo di aerei che dovrebbero servire per la nostra difesa. nostra difesa. Se facessimo un sondaggio tra gli italiani, dubito che meno del 90 per cento approverebbe la linea che stiamo qui proponendo,

visto che l'installazione di queste bombe dovrebbe avvenire alla fine del presente decennio e ancora abbiamo tempo per programmare come dobbiamo attrezzare i nostri aerei, abbiamo tutto il tempo per decidere di non acquisire i requisiti *software* e *hardware* che dovrebbero gestire bombe nucleari a bordo di questi aerei ovvero di

a riformulare la richiesta di non acquisizione dei requisiti *hardware* e *software*, eventualmente cambiandola con un impegno a non installare bombe nucleari su questi aerei a meno che non ci sia un'approvazione esplicita del Parlamento

quindi, sarebbe interesse di tutti i popoli della terra fare degli sforzi e mettere in atto procedure, trattati e impegni per arrivare finalmente al bando di tali armi. L'articolo VI del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, armi nucleari, ratificato dal nostro Paese nel 1975, impegna ciascuna parte a perseguire in buona fede negoziati per definire nel più breve tempo possibile misure effettive che conducano alla cessazione della corsa agli armamenti nucleari e quindi al disarmo nucleare. Secondo il parere della Corte internazionale di giustizia de L'Aja dell'8 luglio 1996, in applicazione del diritto internazionale sono illegittimi la minaccia o l'uso delle armi nucleari. Pur non volendo la Corte esprimersi in merito al caso estremo di legittima autodifesa, viene inoltre chiarito come gli Stati debbano, in ogni caso, rispettare il diritto umanitario internazionale. Ciascuno degli Stati militarmente non nucleari che risulti parte del Trattato di non

l'Italia, in contrasto con tale obbligo e con l'articolo 26 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati

delle armi nucleari, sotto una pressione molto forte proveniente da moltissime organizzazioni a livello internazionale. A votare a favore sono stati 122 Paesi, ma purtroppo tra questi non c'è l'Italia.

soprattutto degli Stati Uniti e della NATO. È chiaro che l'approvazione del trattato non costituisce certamente la risoluzione del problema, anche perché purtroppo l'ONU

alla liberazione del nostro territorio dalle armi nucleari presenti nelle basi e nei porti italiani e quindi a liberare le nostre popolazioni da queste servitù, che non sono semplicemente militari, ma che comportano anche

il Trattato per la messa al bando delle armi nucleari. Signora Presidente, colleghi, siamo passati a parlare delle mozioni sul trattato che rende illegali tutte le armi nucleari al mondo, al mondo, adottato lo scorso venerdì 7 luglio a New York. Io ero personalmente presente e ho seguito tutte le fasi di questa storica approvazione che, dopo i trattati che già tempo fa hanno reso illegali le armi biologiche e chimiche, adesso aggiunge quest'altro tassello verso un progressivo disarmo dell'umanità dichiarando illegali anche le armi nucleari. È un Trattato che è stato approvato da 122 Stati all'ONU e tra questi non ci sono gli Stati della NATO, proprio quelli che sono in possesso di armi nucleari.

in quanto l'articolo 6 del Trattato di non proliferazione nucleare, che dichiarava che ci sarebbe dovuto essere un avvio di trattative per eliminare le armi nucleari già presenti, di fatto non ha funzionato granché:

di aderire a questo Trattato giuridicamente vincolante per vietare le armi nucleari, ai cui lavori l'Italia non ha partecipato, ma visto il grandissimo successo e la decisa approvazione da parte di un così ampio numero di Stati, è ovvio che il cammino è tracciato verso

di chiunque abiti entro un certo raggio dal punto in cui dovessero essere utilizzate. Sicuramente le armi nucleari non svolgono più, anche da quando il mondo è cambiato dopo il crollo del muro di Berlino, alcuna funzione di equilibrio tra potenze, ma costituiscono soltanto un pericolo costante sia di possibile incidente, sia di possibile uso scriteriato da parte del

non necessariamente lo erano rispetto al Trattato di non proliferazione nucleare del 1968. Credo che non si possa non aderire ad una mozione come questa, che allinea l'Italia alla stragrande maggioranza delle potenze e della popolazione mondiale,

Il problema è come si fanno funzionare eventualmente le centrali e come si usa il deterrente nucleare, in questo caso militare. Abbiamo visto che le maggiori potenze hanno sempre utilizzato

le armi nucleari hanno contribuito a mantenere su tutto il pianeta un clima sostanziale di pace. Quello che a noi preoccupa, semmai, è il fatto che si stanno avvicinando al nucleare, mentre altri in parte lo hanno già raggiunto, Paesi che non hanno la nostra cultura di strategia statale o di razionalità completamente avulsi dai criteri occidentali. Dobbiamo anche dire che le motivazioni che hanno spinto noi a entrare nell'Alleanza atlantica e a mantenere mantenere le armi nucleari americane sui nostri territori non sono per nulla venute meno. A maggior ragione, ricordiamo che non ci fu imposto assolutamente nulla, ma furono i Paesi europei a chiedere, anzi a suo tempo a esigere, lo stazionamento nel nel continente europeo delle armi nucleari americane. Circolano dei dubbi sull'affievolimento dell'interesse degli Stati Uniti globale europea. Bene, questa ventilata ipotesi sta già provocando, sia in Germania che in altre Nazioni, un dibattito sull'opportunità di dotarsi di un proprio deterrente nucleare nazionale. Il rischio, pertanto, di un potenziale ritiro di armi nucleari americane in Europa non sarebbe una cosa buona, perché provocherebbe un riarmo nucleare nazionale

Dobbiamo guardare con estrema preoccupazione anche al deteriorarsi della situazione in Estremo Oriente. Parliamo della Corea, che a questo punto spinge un'altra Nazione, e cioè il Giappone, a pensare all'acquisizione di armi nucleari. Non possiamo ritenere che il Giappone, prospiciente alla Corea, dopo una serie di ipotetici attacchi provocatori, possa rimanere in balia del del Governo coreano, che - ahimè - oggi sappiamo da chi e come è orientato e gestito. Un'assenza dell'ombrello nucleare americano provocherebbe

nucleari; di utilizzare la nostra posizione strategica per riuscire a far dialogare le potenze nucleari e a condurle su queste posizioni; di impegnare il nostro Paese a operare nei confronti dei nostri alleati - la Germania per vicinanza e il Giappone per questioni di alleanza atlantica - affinché riflettano sull'opportunità di dotarsi anch'essi di arsenali nucleari.

non c'è dubbio che la proliferazione delle armi nucleari rappresenti ancora oggi una delle maggiori minacce alla pace e alla sicurezza internazionale. Come è noto, il TNP è alla base del sistema internazionale di non proliferazione nucleare e prevede tre obiettivi fondamentali: la non proliferazione nucleare, ovvero la limitazione dei Paesi militarmente nucleari a quelli previsti dal Trattato, che coincidono con i cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza; il disarmo nucleare, in una cornice di sicurezza bilanciata con il relativo impegno dei cinque Paesi in questione; lo sviluppo degli usi pacifici della tecnologia nucleare. Il Trattato è in vigore dal 5 marzo 1970 e la sua implementazione prevede una conferenza di riesame ogni cinque anni. È da poco iniziato il ciclo di riesame destinato a concludersi nel 2020 con lo svolgimento a Vienna, dal 2 al 12 maggio scorso, della prima sessione della conferenza preparatoria. di un Accordo che l'Italia ha ratificato fin dal 1975 e, quindi, di un impegno di lungo periodo per il nostro Paese che, soprattutto per quanto riguarda le politiche di difesa e sicurezza, ha sempre fatto del consolidamento delle istituzioni e degli strumenti multilaterali una delle proprie scelte di fondo irrinunciabili per la tutela della stabilità. Due sono le osservazioni di fondo in merito allo scenario odierno. La prima è che la proliferazione nucleare continua a rappresentare un rischio nel contesto internazionale: abbiamo l'esempio della Corea del Nord, che continua a costituire una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale con l'attivo perseguimento di un programma militare, nucleare e missilistico. La seconda osservazione - come constatiamo ormai da diversi anni - è relativa allo stato di difficoltà delle condizioni di sicurezza nel contesto di oggi e alla nuova fragilità delle relazioni internazionali, che ha determinato una perdita di capacità di *governance* del sistema di sicurezza collettivo,

un confronto compiuto e pienamente consapevole dei temi in discussione non può di certo essere ridotto alle caratteristiche tecniche di un singolo assetto d'arma, come si sostiene in una delle mozioni presentate. Credo che, posta così la questione, sia abbastanza chiaro su quale strada intendiamo proseguire. Siamo per l'adesione delle grandi democrazie a un programma comune per rimettere al centro della propria azione la decisione delle Nazioni Unite, il diritto internazionale e il Trattato di non proliferazione nucleare. Ciò senza ovviamente dimenticare l'ineludibile necessità che tutti gli Stati, gli Stati, incluse le potenze nucleari, si impegnino all'attuazione degli obblighi del Trattato di non proliferazione nucleare in tutti e tre i suoi obiettivi fondamentali, perché gli strumenti multilaterali, oggi più che mai, rappresentano l'unica via per far fronte alle difficoltà e alla complessità di oggi. per quanto riguarda il Trattato di non proliferazione nucleare, è necessario proseguire nella promozione di un approccio progressivo e bilanciato al disarmo nucleare, che tenga conto degli equilibri di sicurezza, in ossequio agli obblighi del Trattato di non proliferazione nucleare, con l'obiettivo ultimo di un mondo privo di armi nucleari.

prova a riflettere attorno alle questioni che sono state già sottolineate dai colleghi e su cui non tornerò. In particolare, vorrei provare a contestualizzare il tema oggetto delle mozioni e, quindi, il Trattato approvato dalla Conferenza dell'ONU appositamente convocata il 7 luglio scorso. Dopo la conclusione del Secondo conflitto mondiale e l'instaurarsi molto veloce della guerra fredda, le armi nucleari hanno rappresentato certamente un elemento di deterrenza e hanno contribuito,

modo la possibilità per cinque Nazioni (le ricordo: Stati Uniti, Russia, Cina, Francia e Regno Unito) di poter mantenere e alimentare un arsenale nucleare. Si sono, poi, aggiunti India, Pakistan, Israele, Corea del Nord

con un forte deterioramento degli equilibri e, conseguentemente, con rischi crescenti, l'ultimo dei quali è certamente l'aggressività in termini nucleari della Corea del Nord. C'è, poi, un secondo elemento che ha mutato il

in alcuni casi, a rendere più facile l'utilizzo delle armi, con le conseguenze negative che ricordiamo che tutti - credo - condividiamo. Con questo spirito abbiamo ripercorso nella mozione i vari passaggi, iniziati il 23 dicembre 2016 con l'approvazione della risoluzione per l'avvio dei negoziati, fino - come già ricordato - all'approvazione il 7 luglio La nostra posizione da questo punto di vista è molto realistica: credo che non possiamo dimenticare l'esistenza di accordi internazionali di difesa NATO e con gli Stati Uniti, che è un elemento che deve essere tenuto in considerazione e, conseguentemente, reso coerente con l'obiettivo, su cui siamo assolutamente d'accordo, di arrivare, in una prospettiva la più breve possibile, al divieto dell'utilizzo delle armi nucleari Da questo punto di vista, il nostro dispositivo - mi avvio alla conclusione per rispettare i tempi - impegna il Governo ad adottare, attraverso la nuova strategia diplomatica, azioni opportune al fine di consentire, nel rispetto degli impegni internazionali già assunti, la sottoscrizione del Trattato giuridicamente vincolante sul divieto delle armi nucleari, approvato a New York il 7 luglio 2017 dalla Conferenza ONU appositamente convocata, dando così seguito alle conseguenti procedure di ratifica dello stesso.

prima di esprimermi nel merito di questa discussione, vorrei evidenziare come l'Assemblea si trovi ad affrontare argomenti importanti quando sarebbe stato auspicabile un approfondimento anche nelle Commissioni di merito, visto inoltre quanto avviato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite dal dicembre 2016, con l'approvazione di una risoluzione che ha disposto l'avvio di negoziati per definire un accordo internazionale «per proibire le armi nucleari e arrivare alla loro totale eliminazione». Indubbiamente, il tema del disarmo e della non proliferazione delle armi porta con sé un carico storico non eludibile, che affonda le proprie radici nella Seconda guerra mondiale, attraverso la corsa agli armamenti della guerra fredda, e arriva a oggi, depositandoci davanti agli occhi una serie di incomprensioni interpretative, non mancando di produrre posizioni politiche talvolta anacronistiche rispetto ai mutati assetti internazionali. Mi permetto di sottolineare che il tema proposto dalla mozione presentata dal collega Cotti è sicuramente meritevole di attenzione, sebbene appartenente a un tema più complesso, quello del sistema d'arma F35, su cui il Parlamento si è più volte trovato a discutere. Ricordando l'audizione del capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, generale di squadra aerea Enzo Vecciarelli, lo scorso 18 maggio, mi sono persuaso che sarebbe stato più utile insistere in quella sede e su questo punto specifico, facendo emergere quali siano le reali capacità del caccia multiruolo. Le mozioni che stiamo discutendo oggi, però, mettono giustamente in luce gli impegni assunti a livello internazionale per difendere quanto contenuto nel trattato di non proliferazione nucleare e, allo stesso tempo, con meritoria razionalità e oggettività, il delicato compito del superamento delle armi nucleari in un contesto geopolitico, come quello attuale, in forte evoluzione. Un chiaro esempio di come si siano disallineati i tradizionali equilibri tra potenze è il programma nucleare e balistico della Corea del Nord, Paese che è uscito dal Trattato di non proliferazione nucleare e costituisce una seria e crescente minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale. Tale circostanza è fermamente condannata dal nostro Paese e rimarcata nella dichiarazione del G7 sulla non proliferazione e il disarmo adottata a Lucca l'11 aprile 2017. Occorre altresì rilevare che, sebbene sia in corso una riduzione del numero complessivo degli armamenti atomici, alcuni Paesi stanno sviluppando nuove capacità tattiche e incrementando i rispettivi arsenali. Mi riferisco a India, Pakistan e Cina. Si deve anche sottolineare che sia Stati Uniti che Russia, che detengono il 93 per cento delle testate, continuano a ritenere gli ordigni nucleari un elemento imprescindibile per i propri piani di sicurezza, tant'è vero che l'amministrazione Obama è passata dal promettere di liberare il mondo dalle armi nucleari all'investire 1.000 miliardi di dollari in trent'anni per ammodernare il proprio complesso nucleare. E si può dire lo stesso anche per la Russia di Putin, con le 7.290 testate e il suo piano decennale per 8 nuovi sottomarini classe Borei, in grado di imbarcare fino a 16 missili Bulava. La Federazione russa ha inoltre deciso di riprendere la produzione del bombardiere supersonico Tupolev Tu-160, con almeno 50 aeromobili da procurarsi a partire dal 2023. Stiamo parlando di sistemi d'arma con capacità balistiche che, per la sola componente subacquea, prevedono una gittata di 10.000 chilometri. Appare chiaro che, se l'obiettivo è quello di un mondo privo di armi nucleari, occorre trovare nuovi strumenti internazionali che superino quelli attuali, basati su un approccio progressivo alla denuclearizzazione. Non sfugge la complessità di una posizione unitaria in un contesto di forti asimmetrie sia sul piano nazionale, che tra i Paesi aderenti al TNP, in quanto vi sono Paesi che detengono armi nucleari, Paesi che le ospitano e Paesi che non fanno parte della Nato. Indubbiamente, è tramontata l'inconsapevolezza del pilota dell'Enola Gay e il timore della proliferazione nucleare, nata con la scissione dell'atomo, ha trovato forza e consistenza in tutti i trattati. È quindi nostro compito mantenere saldo l'impegno a non provocare mai più catastrofi nucleari, con conseguenti danni irreversibili per l'umanità e il pianeta. E l'unico modo per assicurarsi questo risultato è impegnarsi a eliminare radicalmente il rischio. Nel mondo c'è chi accumula ordigni nucleari e li sfoggia come trofei per irretire gli scontri tra potenze, fomentare l'irresponsabilità e cercare *casus belli* adatti allo scontro diretto. È opportuno chiedersi qual è il comportamento più adatto da mantenere, come Paese e come unioni di Stati sotto l'egida comunitaria e di ONU e NATO. Quali sono le strategie da adottare per garantire la pace sullo scacchiere mondiale? Come essere antagonisti in questo contesto di delicati equilibri nucleari? La soluzione non può che essere l'adozione di una nuova strategia diplomatica tesa a consentire, nel rispetto degli impegni internazionali già assunti, la sottoscrizione del Trattato giuridicamente vincolante sul divieto delle armi nucleari, approvato a New York il 7 luglio 2017 dalla Conferenza delle Nazioni Unite.

impegnandoci, a livello nazionale e internazionale, a rafforzare norme che contribuiscano a costruire le fondamenta di un solido futuro di pace. Proprio domenica scorsa è ricorso l'anniversario del primo *test* americano: era il 16 luglio 1945.

non si aveva affatto la consapevolezza del problema delle radiazioni. Ora sappiamo che dal 15 giugno di quest'anno allo scorso venerdì 7 luglio si sono svolti, presso le Nazioni Unite, i negoziati per la stesura e l'adozione del Trattato di messa al bando delle armi nucleari.

Ricordo che quelle nucleari rimangono oggi le uniche armi di distruzione di massa non ancora fuorilegge, nonostante i loro catastrofici impatti ambientali e umanitari, mentre le armi biologiche, chimiche, le mine antiuomo e le bombe a grappolo sono comunque proibite dal diritto internazionale. Oggi nel mondo ci sono almeno 15.000 ordigni, in particolare negli arsenali degli Stati Uniti e della Russia, e sappiamo che altre potenze (Gran Bretagna, Francia, Cina, Israele, India, Pakistan e Corea del Nord) sono dotate di tali strumenti

compatibilmente con l'obiettivo delineato, con gli obblighi assunti in sede di Alleanza atlantica e con l'orientamento degli altri alleati, la possibilità di aderire al trattato giuridicamente vincolante per vietare le armi nucleari, che porti alla loro totale eliminazione, approvato a New York il 7 luglio 2017 dalla conferenza ONU

riguarda l'obiettivo finale, condiviso da tutti, che - come ha già detto il collega Battista - è anche per noi l'eliminazione dell'incubo delle armi nucleari dal nostro pianeta.

sull'obiettivo, che è quello di arrivare in tempi rapidi alla sottoscrizione del Trattato per la messa al bando,

un certo equilibrio. Possiamo perciò dire che le Nazioni che lo hanno utilizzato come deterrente hanno garantito una certa tranquillità e pace a livello internazionale. Quello che più preoccupa sono i Paesi che hanno una cultura militare e nucleare diversa dalla nostra, Paesi che sono arrivati recentemente al nucleare, come il Pakistan, l'India o la Corea del Nord.

completamente dell'area mediterranea ed europea e di ritirare le proprie postazioni. L'Europa tutta dovrebbe prendere una posizione, meditare e pensare alla sicurezza comune in modo diverso. La Germania sta pensando per conto proprio e la Francia vorrebbe imporre un suo modello a livello europeo. Vorrei sapere se dovremo accodarci al fai da te, per cui ognuno deve arrangiarsi, e se l'Europa dovrà seguire un po' il modello francese.

utilizzato da deterrente, il sistema nucleare dal 1945 ad oggi ha dato buoni frutti. Presidente, nella stagione delle facili semplificazioni, in cui tutto deve essere o nero o bianco, dove non esistono le sfumature e non esiste il grigio, bisogna, bisogna, invece, convivere diversamente con i compromessi e, spesso, con gli accordi di mediazione, con la ricerca di equilibri difficili. Nella stagione della memoria cancellata

Stati fuori dall'Unione europea e fuori anche dalla NATO. È la stagione della demagogia dilagante, nella quale si mettono in contrapposizione, nei bilanci degli Stati, le spese militari con le spese per l'istruzione, per la sanità,

per l'esercito, per la militarizzazione, per l'ammodernamento dei propri armamenti. In questa stagione delle semplificazioni, come la semplificazione per la quale talvolta io vedo e sento, in questo Parlamento, un mondo capovolto, l'Italia - e uso un aggettivo inusuale in quest'Aula - è una Nazione buona, una Nazione non aggressiva; non è una Nazione canaglia e malvagia. anche la NATO, per noi, è un'alleanza e una organizzazione difensiva e non aggressiva. Ecco perché, in questa stagione delle semplificazioni, della memoria cancellata e della demagogia, sarebbe certamente incantevole sognare un mondo libero dalle armi e dichiararsi antinucleare e antimilitarista. Invece, la realtà è molto diversa. Il mondo non è fatto solo di anime belle. Nel mondo gli Stati non democratici sono troppi, sono la maggioranza. Il mondo si compone di Nazioni quali la Corea del Nord, la Cina, il Pakistan, la Russia, ma anche l'India, che possiedono armamenti nucleari senza avere il primo vero e unico deterrente al loro uso. Il vero deterrente all'uso dell'arma atomica sono la democrazia, la libertà vera, l'esistenza

proprio negli importanti Stati che detengono l'arma nucleare, ci sono al vertice dittatori, partiti unici e sistemi nei quali gli oppositori e i rappresentanti della stampa vengono arrestati o liquidati. È in questo mondo, e non nel mondo di Alice nel Paese delle meraviglie, che cadono le mozioni che oggi discutiamo e fra poco voteremo. Noi di Area popolare-Centristi per l'Europa siamo favorevoli a quelle mozioni che sostengono il disarmo nucleare con un approccio progressivo, negoziato e controllato; in ogni caso, con un approccio non unilaterale. Essere non unilaterali ha consentito di abbattere il muro di Berlino, di ridurre il numero degli armamenti nucleari tra le due grandi potenze del secolo scorso, di trovare la strada per accordi e trattati di non proliferazione. La deterrenza serve per preservare equilibri, per fortificare la pace e per mantenere e diffondere nel tempo le conquiste occidentali di libertà e democrazia.

Sono però anche le armi che mettono in pericolo la sopravvivenza della specie umana e del Pianeta,

La mozione n. 817 nella sua prima versione avrebbe avuto il nostro voto favorevole. Avendo accettato la riformulazione e, quindi, essendo

e, a maggior ragione, dovremmo occuparci non solo di questioni generali, perché il Trattato avrebbe un effetto benefico anche sul nostro Paese.

una curiosità. A questa associazione, che si è fortemente battuta per l'adozione del Trattato e che di recente ha fatto un appello alla NATO e all'OSCE affinché sostengano il Trattato che bandisce tutte le armi nucleari al mondo, aderiscono 45 parlamentari italiani, tra cui il sottoscritto. Io sono l'unico dell'opposizione

Chiti e Finocchiaro, Granaiola, Pegorer, Mattesini, il capogruppo Zanda, il senatore Zavoli e, persino, il ministro della difesa Pinotti. Aderiscono tutti a questa associazione, che è una di quelle che si è più battuta

datato 1968. Scusate, colleghi, ma è come se ci richiamassimo ai patti di pace siglati dall'impero romano

dare un segnale anche alla nostra popolazione che non vuole armi nucleari sul territorio, figuriamoci quindi se le vuole a bordo dei nostri aerei che volano in cielo.

preliminarmente Forza Italia condivide gli obiettivi individuati dalle mozioni nn. 799 e 801 affinché si persegua un limite nella proliferazione delle armi nucleari. convinti che per raggiungere tale alto scopo sia necessario e fondamentale perseguire un proficuo dialogo nei più alti consessi che coinvolga soprattutto i Paesi che detengono gli arsenali nucleari, ma tutto ciò evidentemente non basta. Tra i Paesi che possiedono armi nucleari vi sono i principali protagonisti della pace siglata dopo la Seconda guerra mondiale, i quali, dalla tragedia nucleare che portò alla rapida conclusione di quel conflitto, trassero comunque l'insegnamento di non utilizzare mai più armi nucleari. Sono naturalmente gli stessi protagonisti della cosiddetta guerra fredda, Stati Uniti e Russia, che hanno utilizzato i propri arsenali per garantire principalmente quella deterrenza che negli anni ha arginato una maggiore proliferazione. *si vis pacem, para bellum* è talmente antica che non ha mai perso la sua attualità. D'altra parte, la cosa più importante rispetto alla presenza nel mondo di armamenti nucleari è che essi, seppur prodotti e immagazzinati, non siano mai utilizzati. Di certo è da condividere l'idea di continuare a lavorare contestualmente per la pace e per un bilanciamento degli arsenali al fine di una loro graduale riduzione. Sarebbe certamente bello un mondo senza armi nucleari, con le grandi potenze impegnate ad utilizzare le risorse economiche per scopi alti e nobili, anziché per costruire ordigni atomici. Tuttavia si illude chi pensa a un mondo senza armi ancora di più chi immagina un pianeta in cui vi siano Paesi pronti a non impiegare una parte del proprio bilancio economico per costruire legittimamente armi. Non vanno poi dimenticati, ai giorni nostri, i cosiddetti Stati canaglia, pericolosamente in grado di produrre armi nucleari di disattendere, oltre i diritti umani più basilari, anche eventuali firme in calce a un qualsiasi trattato di denuclearizzazione. Si rende, quindi, necessaria un'azione di bilanciamento che consenta non una visione manichea tra le forze del bene e quelle del male, ma di contenere le spinte radicali di chi immagini di affrontare i rapporti di potere fra Stati attraverso la minaccia dell'uso o la cessione a terzi di armamenti nucleari. In tal senso siamo certamente favorevoli all'universalizzazione e al rafforzamento del Trattato di non proliferazione, così come riteniamo positiva l'entrata in vigore del Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT). Auspichiamo tuttavia anche la conclusione di un trattato sulla messa al bando del materiale fissile idoneo alla fabbricazione di armi nucleari, il consolidamento e la creazione di zone libere da ordigni atomici. Privo di alcun effetto pratico, viceversa, è il Trattato sul divieto delle armi nucleari votato recentemente all'ONU, opportunamente manchevole del consenso italiano, in quanto sprovvisto di quello delle potenze che possiedono tali ordigni.

In questo non vediamo contrapposizione tra il ruolo degli Stati Uniti e quello della Federazione russa, le due principali potenze nucleari che hanno le più importanti relazioni internazionali ed i maggiori poteri in seno al Consiglio di sicurezza dell'ONU. Paesi impegnati, oltretutto, in maniera preponderante a contenere e fermare il terrorismo che incendia il mondo, continua a devastare il Medio Oriente, e a cui va impedita la possibilità di acquisire ordigni devastanti. Così come, tra i principali attori impegnati a mantenere la pace nel mondo va ricordato che vi sono anche Paesi europei come il Regno Unito, peraltro in fase di uscita dall'Unione, e la Francia, che rimarrà, al momento, l'unico Paese dell'Unione a possedere ordigni atomici,

i propositi della mozione che propone la limitazione all'utilizzo degli F-35 da parte dell'Italia, disattendendo, peraltro, ad impegni già assunti in sede di Alleanza atlantica. L'Italia, come è noto, non dispone di armi nucleari. L'acquisizione degli F-35, che andranno a sostituire macchine a fine vita operativa, per quanto in grado di trasportare armamento nucleare, non vorrà certo significare dotarsi di tali ordigni.

dopo una fase in cui sembrava che il tema del nucleare, in fondo, all'interno del Trattato di non proliferazione nucleare, determinasse una necessità mondiale di riduzione degli armamenti fino a far sparire completamente gli armamenti nucleari. Abbiamo visto che la situazione internazionale si è profondamente modificata dalla fase in cui le due grandi potenze - gli Stati Uniti d'America e l'allora Unione Sovietica - basavano gran parte della deterrenza nell'equilibrio tra le grandi potenze proprio

Si ratificavano, ad esempio, alle Nazioni Unite i diversi Trattati di non proliferazione e sviluppo nucleare, si impegnavano i Paesi a stare all'interno di un certo regime. Con la scomparsa di questa polarizzazione siamo arrivati ad una fase che è, per certi aspetti, più rischiosa che in passato e per questo l'attenzione sullo sviluppo degli armamenti nucleari deve restare molto alta. più rischiosa, perché con la dissoluzione dell'impero sovietico gli armamenti nucleari si sono in parte dispersi in vari Paesi, anche in Paesi la cui stabilità o la cui riconoscibilità democratica è particolarmente dubbia.

Si stanno creando le condizioni per le quali tutti i contenuti del Trattato di non proliferazione, che avevano come pilastro il disarmo e la non proliferazione ed anche l'uso pacifico dell'energia nucleare, vanno rivisitati

della difesa, sia nel Comunicato di Taormina del 26 e 27 maggio. Noi siamo perché il nostro Governo si impegni a perseguire l'obiettivo di un mondo privo di armi nucleari,

l'entrata in vigore del Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT), la conclusione di un Trattato sulla messa al bando del materiale fissile idoneo alla fabbricazione di armi nucleari (FMCT), il consolidamento e la creazione di zone libere da armi nucleari, soprattutto in Medio oriente,

uno schema di lavoro di politica estera e di politica internazionale, a cui tradizionalmente i nostri Governi si sono attenuti all'interno dell'Alleanza atlantica, ma anche delle Nazioni Unite.

mirando solo su qualche tipo di armamento piuttosto che su altri. Tutto questo deve avvenire all'interno di una convenzione che si riesca a realizzare tra i diversi Paesi e sulla quale i diversi Paesi, soprattutto i nostri alleati, debbono poter convenire con noi.

Chiediamo la verifica del numero legale.